Onorevoli colleghi, il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera: «Roma, 15 aprile 2021 Gentile Presidente, informo la Signoria Vostra che con decreti del Presidente della Repubblica in data odierna, adottati su mia proposta, previa approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, della delega di funzioni conferita dal Ministro dello sviluppo economico, è stato attribuito il titolo di Vice Ministro ai Sottosegretari di Stato presso il medesimo Dicastero

nel *week end*. Ricordo che nell'agosto scorso è stato vittima di avvelenamento e che è poi ritornato a gennaio in Russia per scontare la pena di poco più di due anni. C'è però un ricorso pendente presso la Corte dei diritti umani di Strasburgo, in cui il dissidente russo segnala episodi ripetuti di maltrattamento, di privazione del sonno, di malnutrizione e di mancato accesso alle cure mediche. La situazione preoccupa tutte le cancellerie europee e gli Stati Uniti d'America, che sono intervenuti in maniera molto forte, dicendo che, se succede qualcosa ad Alexei Navalny, ci saranno conseguenze. Ieri c'è stato l'incontro fra i Ministri degli affari esteri europei, che non solo hanno espresso preoccupazione, ma hanno chiesto che ci sia l'immediato accesso alle cure mediche. Ricordo che Alexei Navalny è rinchiuso in una colonia penale a 200 chilometri da Mosca, in un reparto ospedaliero, ma

un rischio di violazione dei più elementari diritti umani, come l'accesso alle cure mediche, e per un trattamento umano all'interno delle carceri russe figura che è diventata un simbolo. Ebbene, davanti a un simbolo, sul versante della tutela dei diritti umani, penso che sia giusto che non solo le cancellerie europee e i Ministri degli esteri, come hanno fatto ieri insieme all'alto rappresentante

accedere alle cure, perché finalmente la Russia risponda alla notifica della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, in cui le vengono chieste spiegazioni proprio sulla necessità di dare accesso alle cure, e se non sia necessario liberarlo per permettergli di andare in un ospedale, in una struttura sanitaria di qualità che possa curarlo, tenendo conto del fatto che è stato avvelenato. Pensavo fosse giusto attirare l'attenzione del Parlamento, per poter dare voce anche ai parlamentari e non solo al Governo.

non è tollerabile che un uomo dell'opposizione venga privato della libertà e tenuto in carcere ed ancora meno tollerabile è il fatto che gli si precluda l'esercizio di un diritto primario come quello alla salute.

alla richiesta che si proceda celermente alla tutela della salute di Alexei Navalny. Il fatto che sia stato trasferito nell'ospedale militare non è una garanzia sufficiente. Tra l'altro, siamo anche molto preoccupati del massiccio dispiegamento di truppe russe al confine con l'Ucraina, quindi riteniamo che debba continuare l'impegno delle autorità - *in primis* dell'Unione europea - confermato anche nell'incontro dei Ministri degli affari esteri tenutosi ieri, affinché il dialogo con la Russia continui, ma che questo non precluda la tutela dei diritti, in particolare dell'oppositore Navalny.

attualmente ricoverato nell'ospedale di una colonia penale russa. Per la nostra forza politica, la difesa dei diritti umani è un valore imprescindibile, come la difesa dei diritti civili e delle libertà democratiche. Il dissenso è un valore che non può essere soffocato in alcun modo, sempre e ovunque. Secondo un recente *report* di Amnesty International, sono molti i Paesi in cui le violazioni dei diritti umani sono sistematiche. Purtroppo, questo accade anche in Occidente, nel nostro mondo libero. Cito solo il caso emblematico di Julian Assange, trattato peggio di un dissidente, come un traditore, e ridotto in fin di vita non per una sua forma di protesta, ma per le condizioni di detenzione a cui è stato sottoposto nel Regno Unito. I diritti umani vanno difesi in quanto valore assoluto e non a seconda del Paese in cui vengono violati e soprattutto non devono essere strumentalizzati a scopo politico, tanto più quando questo rischia di aggravare una situazione di tensione già molto preoccupante e pericolosa, come quella che sta montando in Ucraina, dove rischiamo una nuova guerra alle porte d'Europa. Siamo certi che la Farnesina si adopererà nelle sedi competenti per riaffermare l'importanza del rispetto dei diritti umani e dei diritti civili nel mondo, in Russia e ovunque essi vengano violati. La nostra forza politica, il MoVimento 5 Stelle, esprime massima vicinanza a Navalny e a tutti i dissidenti detenuti e ai prigionieri politici che soffrono per portare avanti le loro idee.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, la Camera dei deputati ha approvato lo scorso 31 marzo il disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, esitato in prima lettura da quest'Assemblea il 29 ottobre. 29 ottobre. La 14a Commissione ha proceduto a calendarizzare il testo con tempestività e, una volta ricevuti i prescritti pareri, lo ha approvato senza ulteriori modifiche lo scorso 14 aprile. Faccio presente che non sono stati presentati emendamenti né ordini del giorno, anche perché la Camera ha modificato il testo del Senato in un solo punto, inserendo nell'allegato A la direttiva europea n. 343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. l'allegato A elenca le direttive che il Governo è delegato a recepire, in base all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge, che reca la delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione degli atti dell'Unione europea. Il disegno di legge che abbiamo approvato in Commissione si compone di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 39 direttive europee, inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 16 regolamenti europei. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 18 direttive. Per quanto riguarda l'inserimento nell'allegato A della direttiva n. 343 del 2016 (parliamo di presunzione di innocenza), che ha quale termine di recepimento il 1° aprile 2018, va ricordato che la delega per l'attuazione della direttiva era già stata inserita nella legge n. 163 del 25 ottobre 2017. Tale delega, però, non è stata mai esercitata dal Governo italiano, poiché, a seguito di una ricognizione effettuata, è risultato che il nostro ordinamento interno è già pienamente conforme ai contenuti sostanziali e ai diritti fissati dalla stessa direttiva. Si è deciso pertanto di non procedere al recepimento, informando la Commissione europea prima della scadenza del 1° aprile 2018. La Commissione europea peraltro, nonostante la scadenza del termine, non ha ritenuto di aprire alcuna procedura di infrazione a carico dello Stato italiano per mancato recepimento, né successivamente per violazione della stessa. Va ricordato che la direttiva di cui parlo, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza ed il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, intende tutelare la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie e di polizia e anche il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale. La direttiva si applica a qualsiasi persona indagata o imputata in un procedimento penale e riguarda tutte le fasi di quel procedimento. Corollari della presunzione di innocenza sono i seguenti principi, che gli Stati membri dovranno garantire: l'onere della prova della colpevolezza incombe sulla pubblica accusa; l'indagato ha diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi e tale silenzio non dovrà essere utilizzato contro di lui, né in alcun modo valutato ai fini della commissione del reato; la direttiva riconosce inoltre alla persona indagata o imputata in un procedimento penale il diritto di presenziare al proprio processo; se il principio della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare sono violati, gli Stati devono garantire mezzi di ricorso adeguati. Infine, tenuto conto che i principi affermati dalla direttiva sono già patrimonio dei diritti fondamentali sanciti sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sia dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo, nella direttiva è stata inserita una clausola di non regressione rispetto al consolidamento di tali diritti nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Va anche ricordato che il 31 marzo 2021 la Commissione europea ha pubblicato una relazione sull'attuazione della direttiva nella cui valutazione generale viene evidenziato che la maggior parte degli Stati membri ha adempiuto all'obbligo di recepimento. presenti alcune difficoltà in alcuni Stati membri, riguardanti soprattutto l'ambito di applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva ed il recepimento delle disposizioni relative al divieto di riferimento in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincriminarsi. Il mancato rispetto di tutte le disposizioni influisce negativamente sull'effettività dei diritti da essa previsti. In base alla relazione del 31 marzo, la Commissione europea si riserva il diritto di aprire procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che si dovessero ritenere inadempienti alle prescrizioni della direttiva. Tenuto conto di quanto evidenziato, si è ritenuto quindi di dover confermare il testo approvato dalla Camera dei deputati al fine di permettere l'immediata entrata in vigore della legge di delegazione europea 2019-2020. Voglio aggiungere che in Commissione è stata posta dal senatore Briziarelli una questione con riferimento all'articolo 14 del disegno di legge in materia di sanità animale per evidenziare come il criterio di delega di cui alla lettera andrebbe oltre quanto prescritto dal regolamento n. 429, prevedendo uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica esotica, con pesanti ripercussioni sia sui cittadini, sia sui comparti economici legati a tale attività. In riferimento però a tale tematica, trattandosi di una parte del testo non modificata dalla Camera dei deputati e pertanto non oggetto di esame, abbiamo deciso comunemente che, se del caso, potremmo porre in essere un separato provvedimento legislativo. Ricordo infine che, in riferimento ad alcune delle direttive contenute nel testo, la Commissione europea ha già aperto procedure di infrazione per mancato recepimento dei termini previsti, ed ecco perché abbiamo voluto dare un'accelerazione. Si tratta in particolare delle procedure di infrazione nn. 2021/0121, sulle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri; sul mercato interno dell'energia elettrica; 2021/0058 sugli enti creditizi; 2021/0057, sulle società finanziarie; 2021/0056, sul codice delle comunicazioni elettroniche; sul riciclaggio mediante il diritto penale; 2020/0533, sui servizi di media audiovisivi, e 2020/0070, sull'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema IVA. Siamo quindi in ritardo ed è ora giusto accelerare. Gentile signor Presidente, gentili colleghi, la pandemia da Covid-19 anche nel nostro Paese ha acuito le disparità sociali, scavando un solco ancora più profondo fra chi ancora ha un reddito a fronte di tanti nuovi poveri che la pandemia economica da coronavirus ha generato. Pur consapevole di non poter più integrare il disegno di legge europea che licenziamo oggi mi preme sottolineare la necessità di condividere ufficialmente qui in Aula un emendamento che sarebbe stato adeguato nel contesto di questa legge, ma che presenterò in un prossimo atto legislativo. che ho discusso con molti di voi, riguarda le modalità di arruolamento ai corsi di laurea delle professioni sanitarie ed alle scuole di specializzazione di area medica; esso è correlato all'attuale emergenza pandemica, è limitato nel tempo ed è sperimentale, nell'attesa di una legge di riordino del sistema universitario. Per entrambi gli arruolamenti il test selettivo d'ingresso sarebbe comunque gestito a livello nazionale dal Cinéca e comune per tutti gli atenei, come avviene oggi, ma con graduatorie di merito locali in quanto il candidato concorrerebbe per l'ingresso in un solo ateneo di sua scelta. La gestione centralizzata nazionale del test selettivo sarebbe garanzia di imparzialità ed omogeneità e la meritocrazia sarebbe sempre tutelata, con l'obiettivo di mantenere sempre "alta l'asticella". L'emendamento, il cui testo sarà messo a disposizione dell'Assemblea in una memoria che depositerò al termine dei lavori, consta di due commi. II primo comma è correlato alle modalità di arruolamento ai corsi di laurea delle professioni sanitarie; ha una motivazione squisitamente socio-economica. Infatti, allo stato attuale, con l'impiego di una graduatoria nazionale, l'immatricolazione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie in atenei "fuori sede", ovvero lontano dalla propria residenza, diventa possibile solo alla fascia economica benestante, tagliando fuori una grande fetta di popolazione che oggi, anche a causa della pandemia, ha ridotto notevolmente il proprio reddito, non potendosi permettere quindi gli studi universitari di un figlio fuori sede. delle professioni sanitarie lascerei quindi lo studente libero di partecipare alla selezione nell'ateneo in cui lo desidera, in funzione delle proprie motivazioni e possibilità economiche, garantendo sempre il diritto allo studio. Il secondo comma riguarda le modalità di arruolamento alle scuole di specializzazione di area medica; tale provvedimento ha una motivazione prettamente sanitaria. L'arruolamento oggi avviene utilizzando una graduatoria nazionale che determina la formazione di una popolazione studentesca delle scuole di specializzazione abbastanza variegata in funzione dei loro luoghi di origine, che, se pur molto bello da un punto di vista degli scambi culturali, porta a far sì che, una volta terminato il corso di studi, i neospecialisti facciano rientro nella loro Regione di origine, mettendo in crisi il sistema sanitario regionale dove si sono formati. Con un arruolamento con graduatoria locale sarebbe statisticamente molto più probabile un maggior "regionalismo" nella formazione specialistica post-laurea, che metterebbe "al riparo" i sistemi sanitari regionali, specie in regioni come la Sardegna e la Sicilia, dove insiste anche la problematica dell'insularità. Ciascun medico parteciperebbe al concorso per la scuola di specializzazione con il test nazionale, ma nell'ateneo che preferisce. Al fine di consentire di effettuare il test nazionale per l'ingresso non solo in una scuola, sarebbe utile diversificare i test per specialità e fissarli per gruppi in date differenti, consentendo al candidato di presentarsi fino ad un massimo di tre test selettivi l'anno. Da docente universitario e da medico impegnato in politica, ritengo che le università abbiano una grande responsabilità nel dover supportare il sistema sanitario, specie nella formazione specialistica, e che il diritto allo studio vada sempre e comunque garantito e non possa essere vincolato alle possibilità economiche dei singoli. Testo

del Parlamento europeo, che tratta anche della presunzione di innocenza. Credo sia indispensabile che tutti comprendiamo la reale portata di tale direttiva, in quanto dobbiamo assumere in maniera seria l'impegno a darle attuazione. Essa prevede infatti che «gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o di un imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole». È evidente che ciò costituirebbe un cambio di passo, rispetto a qualche mese fa, quando taluno affermava che in carcere non c'erano innocenti e imperava un clima giustizialista e colpevolista, che spesso sottoponeva alla gogna mediatica una persona per il semplice fatto di essere stata indagata, facendola passare, solo per questo, per un sicuro colpevole.

che il più delle volte vengono esposte soltanto in parte, scorporate in senso accusatorio dal complesso delle intercettazioni medesime o delle conversazioni intercettate. Tutto ciò, ovviamente, senza che la difesa abbia alcuna possibilità di intervento. che ogni anno circa 120.000 persone vengono prosciolte o assolte in primo grado: tutti soggetti i cui nomi sono stati dati in pasto all'opinione pubblica, che quasi sempre non cancella il ricordo del momento del coinvolgimento, ma dimentica facilmente l'assoluzione o il proscioglimento. questi soggetti riusciranno a cancellare il ricordo negativo, a recuperare serenità e credibilità, a ritrovare l'armonia familiare e anche sul luogo di lavoro distrutta dalle inevitabili tensioni, conseguenti al coinvolgimento in un procedimento penale? dunque di un tema attualissimo e di estrema rilevanza. Si pensi, a questo riguardo, a una conferenza stampa che è stata fatta nei giorni scorsi ad Oristano, neppure a conclusione delle indagini, bensì all'avvio delle stesse,

Vogliamo parlare poi della notizia di un avviso di garanzia nei confronti di una stimata funzionaria ministeriale, nota per essere una persona integerrima, cui è stata addebitata un'accusa di corruzione? caso, gli interessi in gioco e gli importi provento della corruzione sono assolutamente incongruenti, cosa che avrebbe dovuto imporre la massima prudenza. La notizia è stata invece data in pasto all'opinione pubblica e la persona non ha resistito all'onta e ha tentato di togliersi la vita, non avendo alcun mezzo a disposizione per giustificarsi, difendersi e affrontare in condizioni di parità quell'accusa. Voglio chiarire che non si vuole mettere in discussione l'operato della magistratura, ma è necessario consentirle di svolgere serenamente la propria attività nel rispetto della Costituzione, che prevede appunto il principio di non colpevolezza sino alla sentenza definitiva. Dunque, il tema che stiamo affrontando ha sicuramente rilevanza estrema. Confidiamo moltissimo nella ministra Cartabia, che ha più volte affermato che il faro del suo operato e della sua azione sarà sempre l'osservanza puntuale della nostra Costituzione. Facciamo in modo che questa direttiva europea trovi piena applicazione nel nostro sistema giudiziario, così da tutelare i soggetti più deboli e porre tutte le parti su un piano di parità che oggi è inesistente. Se, come dobbiamo, daremo corso a questa direttiva, il nostro sistema giudiziario ne trarrà sicuramente rilevanti benefici in tema di equità, di giustizia giusta e di credibilità.

Signor Presidente, torniamo a discutere nell'Aula del Senato della legge di delegazione europea, dopo le modifiche al testo approvato alla Camera dei deputati, con cui è stata inserita un'ulteriore direttiva in materia di presunzione di innocenza nell'allegato A. Nel complesso, gli atti legislativi comunitari cui si fa riferimento sono 50, di cui 11 regolamenti e 39 direttive. In ogni caso, vorrei incentrare questo breve intervento sull'articolo 9 del disegno di legge, che reca i criteri direttivi per il recepimento della direttiva europea n. del 2019, in materia di diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale. L'obiettivo della direttiva è di adeguare il quadro normativo degli Stati membri ai rapidi sviluppi tecnologici che incidono sulle modalità con cui opere e altri materiali sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre emergono costantemente nuovi modelli di *business* e nuovi attori. Dunque, in un contesto generale in continua evoluzione, le nuove norme comunitarie prevedono talune eccezioni e limitazioni al diritto d'autore e ai diritti connessi all'ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, favorendo anche la determinazione di procedure per la concessione delle licenze d'uso, in particolare - ma non solo - per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità *online* di opere audiovisive, in modo da garantire un più ampio accesso ai contenuti e alla creazione di un mercato più equo. La normativa europea va così a incidere su alcuni settori, tra cui la ricerca, l'istruzione e la conservazione del patrimonio culturale, in cui le nuove tecnologie digitali consentono rinnovate modalità di utilizzo, una su tutte l'estrazione di dati, garantendo, da un lato, la necessaria protezione degli interessi degli autori e, dall'altro, le esigenze degli utilizzatori pubblici. Si è andati così verso la risoluzione di situazioni che fino a poco tempo fa erano relegate in un limbo di incertezza giuridica in materia di estrazione di testo e di dati, disponendo un'eccezione obbligatoria per le università e gli altri organismi di ricerca, così come per gli istituti di tutela del patrimonio culturale, al diritto esclusivo di riproduzione in modo da favorire il settore della ricerca scientifica in un'ottica quanto più ampia possibile. Per questo motivo, voglio sottolineare l'importanza del contenuto di cui all'articolo 9 del disegno di legge di delegazione europea, con cui si affida al Governo sia il compito di definire quali siano gli enti inclusi nella nozione di istituti di tutela del patrimonio culturale, nell'accezione più ampia possibile, in modo da favorire l'accesso ai beni in essi custoditi, sia di disciplinare le eccezioni e le limitazioni utili per l'estrazione di testo e di dati, in modo da regolare in via generale l'accesso alle gare e i requisiti dei soggetti pubblici non lucrativi coinvolti, quali università, istituti di istruzione superiore, biblioteche e istituti di ricerca. L'obiettivo di ampliare il novero degli altri enti inclusi tra gli istituti di tutela del patrimonio culturale in relazione all'ambito di applicazione della direttiva è un'esigenza fondamentale. In tal senso, non va dimenticato il contenuto del considerando 13 della direttiva, che espressamente dispone che si dovrebbero inserire in tale elenco le biblioteche accessibili al pubblico e i musei, indipendentemente dal tipo di opere o altri materiali che detengono nelle loro collezioni permanenti, nonché gli archivi e gli istituti per la tutela del patrimonio cinematografico o sonoro. Ancora, secondo il legislatore europeo, vi dovrebbero rientrare anche le biblioteche nazionali e gli archivi nazionali e, per quanto concerne i loro archivi e le loro biblioteche accessibili al pubblico, ne dovrebbero altresì far parte gli istituti d'istruzione, gli organismi di ricerca e gli organismi di radiodiffusione pubblici. Molto spesso l'istruzione e la ricerca scientifica nel nostro Paese, nonostante fossero considerate a parole «settore prioritario», hanno scontato conseguenze disastrose derivanti da politiche di definanziamento e razionalizzazione dei costi e delle spese. In molti documenti economici e programmatici, a fronte di pure dichiarazioni di intenti, in cui questi settori venivano ritenuti essenziali per la ripartenza, le risorse pubbliche stanziate sono state invariate o addirittura in diminuzione. L'attuazione della direttiva del 2019, in tale ottica, può rappresentare uno strumento senza dubbio utile a tale causa, fermo restando che saranno la qualità degli investimenti e le modalità con cui essi saranno supportati, in primo luogo a partire dall'uso delle risorse del *recovery plan*, a definire con quale grado di maturità il nostro Paese saprà affrontare le sfide che riguardano la ricerca scientifica, l'istruzione e la cultura, settore in cui l'impatto delle nuove tecnologie può risultare determinante, soprattutto in un'ottica intergenerazionale.

la legge di delegazione europea che ci apprestiamo ad approvare è uno strumento importante di raccordo tra l'ordinamento europeo e l'ordinamento italiano, attraverso il recepimento di direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione. deve essere vissuta come uno strumento di modernizzazione e semplificazione del nostro ordinamento, per dare certezza e non per creare dubbi e incoerenze interpretative.

2019/1151 sull'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Si tratta di una direttiva che vuole favorire la costituzione *online* delle società e la registrazione di loro succursali, con l'obiettivo chiaro di ridurre i costi, le tempistiche e gli oneri amministrativi, in particolare per le piccole e medie imprese. È chiaro che il recepimento di questa direttiva non potrà rappresentare un passo indietro del nostro ordinamento rispetto alla digitalizzazione del diritto societario rispetto alla necessaria semplificazione e flessibilità nell'utilizzo di strumenti da parte delle *start-up* e delle *start-up* innovative. In questi giorni e nelle ultime settimane è salita la preoccupazione del mondo delle *start-up*, in particolare delle *start-up* innovative, rispetto alla possibilità che ci sia un passo indietro. In verità, molte di queste legittime preoccupazioni sono legate a una sentenza del Consiglio di Stato che ha cancellato il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio 2016. È vero che, da oggi e fino a nuovi interventi legislativi, le *start-up* italiane non potranno costituirsi gratuitamente *online.* Ma questo non ha niente a che fare con il disegno di legge che stiamo discutendo e non potrebbe essere altrimenti, essendo una delega. Gli effetti che vediamo e le preoccupazioni che registriamo sono legati alla sentenza del Consiglio di Stato sul decreto ministeriale del 2016. Anzi, l'attuazione dei principi e dei criteri di delega che stiamo per approvare

a responsabilità limitata semplificate, con sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, attraverso due strumenti e lasciando flessibilità nell'utilizzo di questi strumenti agli operatori economici, come è ormai pratica

la videoconferenza e la sottoscrizione da remoto dell'atto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. La seconda possibilità prevede procedure telematiche che, previa identificazione elettronica del richiedente, consentano l'utilizzo di modelli *standard* predefiniti e validati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero della giustizia, da sottoscrivere sempre con firma digitale o altro tipo di forma elettronica qualificata. È opportuno lasciare, quindi, flessibilità negli strumenti di nascita delle nostre imprese, delle *start-up* e delle *start-up* innovative riducendo oneri amministrativi impropri e costi burocratici che non servono se la strada che vogliamo continuare a perseguire è quella di una semplificazione e digitalizzazione del nostro diritto societario. Fermi restando gli Fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione della direttiva dell'Unione, devono essere assicurati i controlli richiesti dall'articolo 10 della stessa direttiva conferendo ai conservatori del registro delle imprese uno specifico potere di controllo amministrativo. Non avrebbe senso recepire la legge di delegazione e la direttiva che la legge di delegazione recepisce facendo fare un passo indietro al percorso di digitalizzazione e semplificazione del nostro diritto societario. Ma questo è perfettamente nei perimetri che il Governo potrà agire e mi auguro che la delega venga esercitata recependo tali principi e rimediando al passo indietro che il superamento del decreto ministeriale del 2016, ad opera del Consiglio di Stato, rischia di farci fare togliendo certezza e ponendo oneri impropri al mondo delle *start-up* e delle *start-up,* innovative della cui vitalità avremo un grande bisogno rispetto alle sfide della nostra economia nei prossimi mesi e anni.

ha già anticipato che sarei intervenuto relativamente al solo articolo 14 della legge di delegazione europea e, in particolare, la posizione della Lega è chiarissima. Proprio questa mattina Matteo Salvini, insieme al collega Campari, ha presentato un disegno di legge a tutela degli animali. Noi siamo per la difesa degli animali, ma non possiamo accettare che con la scusa - e lo dico chiaramente per l'articolo 14 - di tutelare la salute

da imparare da nessuno a livello nazionale e abbiamo aderito già dal 1975 alla Convenzione di Washington per la tutela delle specie protette animali e vegetali.

solo per quest'anno. Un intero comparto fatto di produttori di gabbie, di produttori di mangime, di veterinari specializzati rischia di essere messo in ginocchio non per il recepimento di una disposizione europea (come hanno fatto tutti i Paesi), ma perché, come sempre, noi ci imponiamo qualcosa di più e troviamo la scusa per una battaglia ideologica, per creare un danno a milioni di italiani che hanno in casa un animale d'affezione - non vedo perché, oltre al gatto e al cane, non si anche un altro animale - e per danneggiare un comparto che conta decine di migliaia di addetti e di posti di lavoro. La richiesta che abbiamo avanzato in Commissione, trovando accoglimento da parte del Presidente e dei colleghi, è stata di fare un approfondimento. Preso atto che è impossibile bloccare l'intera

che di fatto non solo non aggiunge nulla in termini di sicurezza per la salute - ben vengano i controlli e la repressione dei fenomeni e delle azioni illecite - ma distrugge un comparto e addirittura potenzialmente

gentili senatrici, il 14 febbraio dello scorso anno il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge di delegazione europea che avvia la procedura di integrazione nell'ordinamento italiano di importanti direttive comunitarie, chiudendo tra l'altro diverse procedure di infrazione nei confronti dell'Italia e risparmiando così denaro pubblico per le relative sanzioni. Oggi, con l'approvazione in terza lettura di questo provvedimento, mettiamo un punto fermo all'importante lavoro svolto in questi mesi alla Camera dei deputati e al Senato. Il Parlamento ha migliorato il testo iniziale, con la consapevolezza del ruolo centrale ricoperto dal nostro Paese in Europa e soprattutto alla luce del ruolo che sta ricoprendo l'Europa nelle more dell'emergenza Covid-19. Il provvedimento che oggi voteremo è di buon auspicio anche per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, perché rappresenta il pilastro su cui si poggerà l'Italia del futuro. È una dotazione importantissima, che, ottenuta da Bruxelles, rappresenta un vero e proprio *new deal* da cui ripartire; si gettano così le basi per i prossimi decenni. Pertanto l'Italia ha il dovere, ancora una volta, di assolvere agli impegni chiesti dall'Europa con responsabilità e solidale collaborazione. Passando al profilo tecnico di questo disegno di legge, possiamo dire che è stato approvato in prima lettura dal Senato il 29 ottobre 2020 e in seconda lettura dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2021. marzo 2021. La Camera ha modificato solamente l'elenco delle direttive, portando a 39 il numero degli atti da recepire nel nostro ordinamento. In particolare, è stata inserita la direttiva (UE) 2016/343, relativa al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Il testo, composto da 29 articoli, reca disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 39 direttive europee e l'adeguamento della normativa nazionale a 17 regolamenti europei. L'approvazione di questa legge consentirà al nostro Paese di fare grandi passi in avanti nell'ambito di due temi che ci stanno molto a cuore: la transizione ecologica e la transizione digitale. A questo proposito, è importante dire che, proprio grazie alla volontà e all'intuizione del MoVimento 5 Stelle, abbiamo dotato il nostro Paese, per la prima volta, di un Ministero della transizione ecologica. Il tema ambientale e della transizione ecologica, che ci ha visto sempre in prima linea, è affrontato in modo particolare da tre articoli: l'articolo 5, l'articolo 12 e l'articolo 22... *(Brusio)*. PRESIDENTE. Mi scusi,

rinnovabili e, infine, la riduzione dell'incidenza di specifici prodotti di plastica sull'ambiente. In materia ambientale - ad esempio - aumenteranno le semplificazioni che consentiranno la diffusione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche e avremo importanti disposizioni per la lotta all'inquinamento delle plastiche, e questo anche attraverso la messa al bando di prodotti monouso, che non sono solo posate, piatti e cannucce - come già previsto nelle direttive europee ma anche bicchieri e ciò grazie ad un emendamento *ad hoc*. Le plastiche biodegradabili, poi, potranno essere utilizzate per i prodotti monouso, quando non siano disponibili alternative riutilizzabili. Infine, è previsto l'avvio di sperimentazioni per un graduale passaggio a un sistema di dispacciamento i cui modelli sono già diffusi in Europa, con l'obiettivo di promuovere un ruolo più attivo dei gestori della rete di distribuzione. Il presente testo di legge delega anche il Governo a riordinare la normativa in materia di autoconsumo, al fine di favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, l'installazione di impianti di produzione di energia negli edifici esistenti e l'individuazione di incentivi volti alla costituzione delle comunità di energie In questo modo l'Unione europea impone agli Stati membri di predisporre un quadro favorevole alla promozione e all'agevolazione dello sviluppo dell'autoconsumo, anche in forma collettiva. L'attivazione, infatti, dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili sono una realtà che - lo voglio sottolineare - l'Italia ha anticipato e precorso grazie al MoVimento 5 Stelle, con un provvedimento apposito approvato oltre un anno fa. Pertanto, grazie al potenziamento di questi strumenti, noi saremo in grado di diminuire il fabbisogno nazionale di energia e le conseguenti emissioni inquinanti, creare nuovi posti di lavoro per le piccole e medie imprese italiane del settore e ridurre il costo delle bollette per i condomini e le abitazioni. Questo è un tema cruciale, se consideriamo che 20 milioni di italiani che vivono all'interno dei condomini sprecano più della metà delle loro bollette. Relativamente invece alla transizione digitale, da sempre riteniamo fondamentale rafforzare il riferimento a tutte le tecnologie che possono garantire l'accelerazione del nostro Paese nella realizzazione di una copertura a banda ultralarga. In particolare, l'articolo 4 della legge dispone criteri e princìpi direttivi per l'attuazione della direttiva europea che disciplina il codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Questo codice ricomprende quattro preesistenti direttive in materia di telecomunicazioni e definisce sia un quadro aggiornato della disciplina delle reti, sia i compiti delle Autorità nazionali di regolamentazione, in vista dello sviluppo delle reti 5G. Pertanto, con il recepimento di questo codice, l'Italia farà un passo in avanti verso l'ammodernamento digitale del nostro Paese; getterà le basi per il rinnovamento della rete e favorirà le infrastrutture adeguate a soddisfare il bisogno di connettività di famiglie e imprese, soprattutto nelle cosiddette aree bianche del Paese, fortemente localizzate nel Mezzogiorno e nelle zone interne. E sottolineo che questo è un obiettivo cruciale, se consideriamo le difficoltà incontrate durante il primo *lockdown* da milioni di cittadini a causa dell'assenza di una connessione adeguata allo svolgimento dello *smart working* e della didattica a distanza. Infine, è importante citare anche una direttiva fondamentale per la tutela del *made in Italy* agroalimentare, cioè quella relativa al contrasto di pratiche commerciali sleali. A vigilare su questa materia sarà l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari. L'Ispettorato, che è presente in maniera capillare sul territorio, ha già mostrato nel tempo la sua capacità di prevenzione e contrasto dei reati in questo settore. Con questa direttiva avrà la possibilità di avvalersi del supporto del Comando per la tutela agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. onorevoli colleghi, dopo i ritardi dovuti al rallentamento dei lavori parlamentari a causa della pandemia e della crisi di Governo, finalmente il Senato oggi darà il via libera definitivo a questa legge di delegazione europea. lo farà anche grazie al voto favorevole del MoVimento 5 Stelle, nella consapevolezza che oggi contribuiamo a fortificare il ponte che collega il nostro Paese con l'Unione europea e, soprattutto, con tutti gli altri Stati membri.

Signor Presidente, ho chiesto di intervenire perché è questa l'occasione per ricordare alcuni problemi che riguardano il nostro Paese, la garanzia dei rapporti tra cittadini alcune garanzie previste dalla nostra Costituzione, anche se è stato introdotto come allegato alla Camera il richiamo alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare nel processo nei Tutto questo si basa su due principi forti della nostra Costituzione. Il primo principio, riguardante la presunzione di non colpevolezza,

nessuno può essere ritenuto colpevole o additato come tale anche se rinviato a giudizio. dall'articolo 16 all'articolo 21 della direttiva esplicitano questo concetto: gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai *media*, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o gli imputati come colpevoli fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata,

la necessaria conseguenza e correlazione del principio di non colpevolezza. Non ci può essere un principio di non colpevolezza se non c'è un giudice terzo e imparziale: è questa la logica. Al contrario, nel nostro sistema abbiamo delle trasmissioni televisive che rappresentano una una celebrazione di un processo per così dire di massa, secondo un modello estraneo alla nostra cultura giuridica e sociale. Badate: nel momento in cui fossero la piazza

principi. Credo che una delle prime regole che il giudice deve imparare nel nostro Paese sia la sua terzietà. Che cosa vuol dire? Se sei giudice della famiglia, devi dimenticare il modello familiare in cui credi. Devi poter sviluppare una capacità di estraneità alla vicenda processuale in modo tale da avere la capacità di delimitare le vicende le vicende di quella famiglia e applicare i principi costituzionali, ma mai con l'intento di interferire in quella famiglia. Così, nel penale o in qualsiasi altro campo, un giudice che pensa di modellare la sua azione al suo credo alle sue convinzioni è fuori dal modello costituzionale: non è un giudice. Il principio di terzietà,

Solo questa è la garanzia del nostro sistema. Noi abbiamo invece il processo mediatico, basato sulla non conoscenza dei fatti. Mi è capitato nella vita, almeno in quattro processi di Mani pulite, di avere una cognizione di certezze matematiche su prove e altri elementi ed avere invece una rappresentazione televisiva completamente distonica. distonica. Presidente, la mia conclusione è che noi abbiamo le regole, ma dobbiamo non solo pretendere

con me e con il Governo la necessità di accelerare. Abbiamo la necessità di chiudere questo procedimento legislativo e mi auguro che con il voto di oggi si possa porre rimedio a tutta una serie di

a ringraziare la 14a Commissione, il presidente Stefano e tutti i commissari per l'ottimo lavoro svolto, perché non solo noi adesso andiamo a recepire il passaggio di proposta della Camera, ma il grosso del lavoro è stato fatto proprio dalla 14a Commissione del ci tengo a fare i dovuti ringraziamenti e - se mi permettete - anche a ringraziare la già sottosegretario Laura Agea, visto che è stata lei a lavorare molto per questa legge di delegazione. Questa è una legge di delegazione che - come diceva la senatrice Ricciardi - costruisce una base per il PNRR e non è un caso che tra le 39 direttive ce ne sono alcune

il codice delle comunicazioni elettroniche, che è cruciale per lo sviluppo della banda larga, proprio per quello che dovremmo fare nel PNRR; le fonti rinnovabili e le direttive sui servizi media-audiovisivi.

su cui l'esercizio e la delega con il Ministero della giustizia lavoreranno intensamente. Vorrei rispondere anche al senatore Doria, per quanto riguarda la proposta che non entra in questa legge di delegazione, ma nella prossima, anche nel passaggio sulla legge europea, e al senatore Briziarelli, per quanto riguarda l'esercizio della delega, perché è evidente che, una volta approvato, avremo due tre mesi con i Ministeri competenti per porre rimedio anche a una lettura appropriata. Lo stesso vale per quanto riguarda l'intervento del senatore Nannicini, che ovviamente sottolineava il punto centrale delle *start-up* e che nell'esercizio della delega anche la costituzione delle società più giovani e più innovative deve vedere

e darci appuntamento già alla prossima settimana per la legge europea e anche per la nuova legge di delegazione, continuando questo lavoro sulla riduzione delle infrazioni per il nostro Paese. Tengo anche a dire che il lavoro fatto all'inizio di quest'anno colloca l'Italia tra i Paesi che stanno riducendo di più e con più velocità le infrazioni, ma sono sicuro che questo Parlamento, con la sua attenzione e con la sua capacità, riuscirà a dare uno stimolo ancora maggiore.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, che ha introdotto una integrazione all'allegato A richiamato dal comma 1 dell'articolo medesimo. Indìco la votazione

Senato approva**. *(v. Allegato B)*. Gli articoli da 2 a 29 sono identici agli articoli del testo approvato dal Senato e non saranno pertanto posti in votazione.

Signor Presidente, siamo chiamati a votare l'unica modifica apportata dalla Camera dei deputati in data 31 marzo al disegno di legge di delegazione europea 2019-2020, già approvato in prima lettura dal Senato nell'ottobre scorso; modifica con la quale è stata inserita una nuova direttiva - come già è stato ricordato - portando a 39 il numero degli atti europei a cui siamo chiamati a dare attuazione. Si tratta della direttiva n. 343 del 2016 in materia di giustizia sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Il termine di recepimento della direttiva era fissato nell'aprile del 2018. Si ricorda, più in generale, che il disegno di legge di delegazione europea consta di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 39 direttive e l'adeguamento dell'ordinamento interno a 16 regolamenti europei; una legge complessa, che ha visto svolgere un gran lavoro da parte della 14a Commissione su materie importanti, dai diritti audiovisivi alle fonti di energia rinnovabile, ambiente, concorrenza e mercato interno, cybersicurezza e anche in materia bancaria e creditizia. In particolare, tuttavia, la direttiva n. 343 del 2016, introdotta con la modifica all'articolo 1, intende tutelare la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie e di polizia e in tutte le fasi del processo, nonché il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale. Corollario della presunzione d'innocenza sono pertanto i seguenti principi che gli Stati dovranno garantire: l'onere della prova della colpevolezza incombe sulla pubblica accusa; l'indagato ha diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi e tale silenzio non dovrà essere utilizzato contro di lui né in alcun modo valutato ai fini della commissione del reato. È bene ricordare che i principi afferenti alla direttiva sono già patrimonio dei diritti fondamentali europei sanciti sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sia dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo peraltro in perfetta aderenza ai principi costituzionali, *ex* articolo 27 della nostra Costituzione, nonché al principio del giusto processo, di cui Tuttavia - ed è questa la parziale novità - il principio europeo della presunzione d'innocenza sembra voler estendere tale diritto per chiedere agli Stati membri di adottare misure al fine di garantire che, nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità procedenti, non ci si riferisca mai in alcun modo alla persona come colpevole, al fine di garantire altresì che le persone indagate o imputate non siano presentate mai come colpevoli in tribunale o in pubblico, per esempio attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica, salvo naturalmente che tali misure non siano necessarie per garantire sicurezza o evitare la fuga. dunque, di una visione di maggior garanzia che potrebbe richiedere peraltro un'azione piuttosto culturale oltre che di richiamo giuridico contro ogni tipo di processo mediatico. La proposta si iscrive nell'ambito delle misure di attuazione del programma di Stoccolma, adottato già nel 2009, che aveva invitato la Commissione a presentare misure volte a rafforzare i diritti dell'indagato o dell'imputato stabilendo norme comuni agli Stati membri. Inoltre, in merito, fino alla direttiva in commento era intervenuta una serie di altre direttive: ricordiamo nel 2010 la direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione; nel 2012 la direttiva sul diritto all'informazione nei procedimenti penali e nel 2013 la direttiva sul diritto ad avvalersi di un difensore anche nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, peraltro già attuata con decreto legislativo del 2016. Le disposizioni della proposta sono da ritenersi conformi, pertanto, all'interesse nazionale, in quanto tese a realizzare il diritto del giusto processo con un sistema di garanzie minime verso una progressiva armonizzazione europea delle fattispecie, che si pone alla base della fiducia reciproca e del riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri. Si tratta, dunque, di un passo ulteriore molto importante verso l'integrazione europea anche in materia di giurisdizione. Per tali motivi dichiaro il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI di legge di delegazione europea 2019-2020, così come modificato dalla Camera

e questo è già indicativo di quanto il percorso del disegno di legge in esame sia stato accidentato. Ancora più indicativo, però, è quanto accaduto nelle scorse votazioni tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica.

pensate un po' - presentato a gennaio 2020, cioè in data antecedente al diffondersi dell'epidemia da Covid-19 e, quindi, ovviamente il documento non faceva alcun cenno alla crisi innescatasi a seguito della pandemia.

il Patto di stabilità); c'era il divieto di erogare aiuti di Stato, anch'esso sospeso. È stato perfino sospeso per un periodo il Trattato di Schengen che prevede la libera circolazione delle persone, uno dei pilastri su cui è stata costruita l'Unione europea, che è stato messo da parte per far fronte alla pandemia che stiamo vivendo anche in questi giorni. E noi abbiamo avuto il coraggio di votare un documento in cui tutto ciò era clamorosamente assente oggi siamo qui di nuovo, in quest'Aula, a discuterne in terza lettura, una perdita di tempo francamente inutile in un contesto europeo dove, ancora una volta, le regole sembrano essere chiare ma non esattamente uguali per tutti. La Germania infatti, ancora una volta, fa sentire forte la sua voce. Lo aveva già fatto lo scorso anno, quando si era posta il problema della legittimità del *quantitative easing*, quando lo scorso 5 maggio la Corte costituzionale tedesca aveva espresso seri dubbi di legittimità su questo strumento. Voglio ricordare che tale strumento prevede l'acquisto di titoli di Stato dei Paesi membri dell'eurozona da parte della Banca centrale europea. Chiaramente la BCE ha fornito spiegazioni che sono state accettate dal Governo tedesco e la Bundesbank potrà continuare a sostenere questo tipo di strumento. Nell'occasione è bene ricordare come la cancelliera Merkel abbia dichiarato chiaramente di volersi attenere alle decisioni della Corte costituzionale tedesca. Ovviamente, queste dichiarazioni della Merkel costituiscono un importante precedente che però non è il solo. solo. Infatti poco meno di un mese fa abbiamo assistito ad un altro *stop* da parte della Germania, questa volta sul *recovery plan;* uno stop tedesco di fronte a un piano europeo molto importante,

Il problema sollevato dai tedeschi è sul debito condiviso previsto dal Next generation EU, di cui beneficia anche la Germania; un debito condiviso dagli Stati dell'Unione che viene ripagato dagli stessi Stati attraverso il bilancio europeo e dopo un anno di discussioni e di trattative dobbiamo registrare che è la Germania della cancelliera Merkel, lo Stato di maggior peso dell'Unione europea, che sta ponendo delle difficoltà. E ora, su questo incredibile *stop* tedesco al *recovery fund*, ci aspettiamo che il Governo e la stessa maggioranza si pronuncino condannando l'atteggiamento della Germania che ogni volta sente il bisogno di ricordare al resto d'Europa che decide tutto lei e che tutti devono sottostare alle sue prese di posizione, anche perché, forse è bene anche qui ricordarlo, in linea strettamente teorica la bocciatura tedesca del Piano farebbe crollare tutta l'impalcatura dello stesso e dovremmo dire definitivamente addio al *recovery* con tutte le conseguenze che ne deriverebbero. Dunque secondo noi di Fratelli d'Italia, vi è una questione di principio per la quale la Germania, ovvero il principale stato dell'Unione europea, dichiara ufficialmente che il suo ordinamento è sovraordinato rispetto alle leggi europee. Quindi non si può certo stare in un consesso in cui le regole stabilite valgono per tutti, ma non per uno dei partecipanti, che decide di fare come meglio crede. noi è una battaglia di dignità nazionale, una battaglia per il rispetto della nostra Costituzione, una battaglia per l'affermazione della sovranità nazionale ed è una battaglia che Fratelli d'Italia conduce da sempre in ogni sede, e che il nostro *leader* nazionale, Giorgia Meloni, ha formalizzato alla Camera con una proposta di legge. In queste settimane, come tutti sapete, abbiamo impegnato il Parlamento con il Piano nazionale di ripresa e resilienza; un piano che abbiamo detto essere superato e obsoleto, già bocciato dall'Europa e che non sarà quello che il Governo presenterà a fine mese che sarà, invece, un Piano nazionale di ripresa e resilienza

a Bruxelles. Peccato che proprio ieri dall'Europa ci hanno fatto sapere che non è fondamentale che il Piano nazionale di ripresa e resilienza venga consegnato entro fine aprile, quanto invece è fondamentale la qualità di questo Piano e che qualche giorno in più non sarebbe certamente un problema per l'Europa. Allora, Presidente, prendiamoci questo tempo in più che serve, facciamo lavorare il Parlamento su un Piano che impegnerà le future generazioni. Vogliamo lanciare ancora un *input*, come ha fatto ieri il nostro presidente Giorgia Meloni nell'incontro avuto con il presidente Draghi, che ha ereditato questo Piano dal precedente Governo e non possiamo fargliene una colpa; però, questo sì, Presidente, vogliamo invitare il nuovo Governo a rispettare la dignità del nostro Paese e del Parlamento, che deve assumere un ruolo baricentrico - come sempre diciamo

aspettandoci che da domani il Parlamento torni ad essere centrale e torni a rappresentare degnamente l'Italia e gli italiani.

sulla quale abbiamo interloquito con tantissimi attori interessati alle direttive. Oggi finalmente diamo risposta ad un tema cruciale: il diritto d'autore. Credo che l'Italia sarà con il voto di oggi il secondo Paese dell'Unione europea a recepire la direttiva sul *copyright*. Una norma di civiltà; gli autori producono cultura e la cultura è il seme della democrazia, della tolleranza, dell'autonomia critica, della responsabile consapevolezza. Come ci ricorda spesso il grande Giulio Rapetti, in arte Mogol, il diritto ad essere remunerati per il proprio lavoro è un diritto basilare e inviolabile.

chiedersi perché del lavoro di circa 90.000 autori ed editori, molti dei quali giovani e al di sotto dei trenta anni, debbano beneficiare gratuitamente i giganti del *web*, che realizzano profitti enormi grazie all'arte e alla creatività di cantanti, scrittori, poeti e attori italiani ed europei. Il lavoro di chi crea sarà un buon lavoro solo se protetto e remunerato. Accanto a questa risposta storica,

inoltre un principio importante: le direttive europee saranno attuate tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia, soprattutto per ciò che riguarda le imprese. Vorrei concludere il mio intervento con una considerazione politica più ampia: bene dunque l'Europa per le direttive che noi oggi recepiamo, bene le nostre due Camere per il lavoro anche lungo, ma intenso che hanno svolto, bene l'Europa sulla sospensione del Patto di stabilità, bene l'Europa sul *recovery plan*, bene l'Europa sugli eurobond*;* devo dire con onestà meno bene devo dire l'Europa sui vaccini. La pandemia avrebbe dovuto inaugurare una nuova stagione globale di cooperazione, invece ha accentuato la competizione geopolitica e il vaccino è diventato la nuova arma nucleare di una nuova guerra per l'egemonia. In questa guerra l'Europa sembra,

è il tema decisivo, senza la cui soluzione tutti saremo più deboli e più soli.

A onor del vero, per quanto riguarda l'inserimento nell'allegato A della direttiva, che aveva come termine di recepimento il 1° aprile 2018,

nonostante fosse scaduto il termine, non aveva ritenuto di aprire alcuna procedura di infrazione. Dico questo per evidenziare che forse avremmo

rafforzato alcuni aspetti relativi alla presunzione d'innocenza e al diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali e tutto quello che va nel senso di affermare i diritti dei cittadini e il garantismo certamente ci vede consenzienti. disegno di legge di delegazione non è stato modificato rispetto al lavoro che è stato fatto dal Senato ormai qualche tempo fa e dunque, nel confermare il nostro voto favorevole, vorrei richiamare alcune questioni questioni molto importanti, che sono presenti all'interno della legge di delegazione europea. Del fronte dell'occupazione si è detto,

Anche nel campo della formazione e della cultura, tra le direttive che il Governo è delegato a recepire, ve ne sono alcune molto importanti: dalla direttiva 2018/1808 2018/1808 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative per quanto riguarda la fornitura di servizi di media audiovisivi all'intervento sui diritti d'autore.

il percorso verso la transizione energetica, i nuovi obiettivi che l'Europa si è data di riduzione delle emissioni, anche in vista del traguardo della neutralità climatica da conseguire nel 2050. Ci sono quindi in questo testo di delegazione molti

stato licenziato dal Senato erano stati approvati una serie di emendamenti anche sul fronte delle rinnovabili, che sono molto importanti e che anzi riteniamo fondamentali per quanto riguarda la questione delle comunità energetiche, dell'auto dispacciamento e dell'autoconsumo. Insomma, una serie di misure che ci aiutano molto nel percorso della transizione verde.

già dal 1° gennaio 2023, anticipando quindi di un anno la direttiva che ne prevede la graduale esclusione tra il 2024 e il 2030, sulla scia di quanto stanno facendo altri Paesi europei, come la Francia, e - credo - facendo così un lavoro molto importante proprio per l'equilibrio del pianeta.

che il Parlamento cede al Governo per adeguare l'impianto normativo alle nuove disposizioni comunitarie. Anche quest'anno sono davvero tante le aree in cui si interviene, come ad esempio la salute, l'ambiente, la cybersicurezza, la finanza, la giustizia: milioni di nostri concittadini, quindi, dovranno avere a che fare con queste nuove norme. L'approvazione del disegno di legge, dunque, è fondamentale per molti evidenti motivi. In primo luogo, è indispensabile per scongiurare il rischio di procedure di infrazione, situazione in cui invece cadiamo spesso e che comporta costi enormi e lunghi contenziosi al nostro Paese. Va detto infatti che troppo spesso la poca attenzione dedicata proprio a questo provvedimento ha comportato per l'Italia conseguenze spiacevoli a livello europeo, il che non è mai un bene sotto vari punti di vista, di costi ma anche di credibilità. Inoltre, approvare questo disegno di legge significa assicurare maggiori tutele e garanzie ai nostri cittadini. Le norme europee, infatti, non impongono solo vincoli, limiti e restrizioni; le regole dell'Unione europea assicurano, anzi, soprattutto diritti, libertà, opportunità per i nostri connazionali. Non rispettare le regole europee o non recepirle correttamente non significa recuperare sovranità; piuttosto significa penalizzare le nostre aziende e i nostri lavoratori e indebolire il nostro Paese rispetto ad altri Stati. Il provvedimento di oggi, quindi, non ha un semplice carattere tecnico o burocratico, ma si occupa di temi concreti ed estremamente innovativi e importanti, con cui tutti dovremmo confrontarci nel nostro futuro quotidiano. È anche l'esatta misura di quanto l'Europa e i suoi Stati membri debbano collaborare concretamente affinché lo sviluppo comunitario sia reale e ampio, con una visione di lungo raggio, che consenta al progetto europeo di trovare sostanza e definitivo compimento. proprio la legge di delegazione europea ci è, quindi, chiaro che lo scopo principale dell'Unione è quello di creare percorsi comunitari che aiutino tutti gli Stati a progredire insieme sulla strada dello sviluppo economico, sociale e culturale, con coesione ed equità. Quando qualcosa si ingolfa, non direi che è colpa dell'Europa, ma dell'uso che i singoli Stati fanno degli strumenti che l'Europa mette loro a disposizione. Con il programma Next generation EU l'Europa ha l'ambizione di trasformare le macerie lasciate dal Covid-19 in una grande opportunità, per ricostruire un continente più competitivo e più efficiente, più moderno e più *green*; un'Europa dei diritti, un'area di libertà economica e sociale. È veramente un'occasione unica, un livello di maturazione comunitaria cui non eravamo quasi più abituati. Ma l'Europa non è un'entità astratta che lavora per conto proprio: serve la nostra collaborazione. La pandemia ha ampiamente dimostrato come i Paesi membri siano totalmente interdipendenti tra loro. A noi quindi il compito di riannodare i fili di un dialogo sempre più stretto con i nostri *partner* europei, per provare a essere ogni giorno che passa più incisivi nella costruzione delle regole comuni, tutelando anche al meglio i nostri interessi. Per farlo è necessario che le direttive che recepiamo oggi, così come i programmi che pensiamo di porre in essere domani, abbiano poi un riscontro concreto e attento nella legislazione nazionale. Spesso, invece, pur approvando provvedimenti che recepiscono le regole europee, noi le interpretiamo male, facendoci del male da soli. Un esempio su tutti lo ha ricordato oggi in un articolo il collega Cangini: il codice degli appalti. Il codice degli appalti, che nasceva dal recepimento della direttiva europea sui lavori pubblici, ci ha visti protagonisti di un richiamo formale da parte dell'Unione stessa per la sua incongruenza con le regole europee, interpretate in maniera eccessivamente restrittiva, fino al punto di diventare ingessatura al nostro sviluppo invece che strumento di uno sviluppo più corretto. Nella complessità del provvedimento oggi al nostro esame vi sono, poi, molti punti fondamentali da valutare con attenzione, in un'ottica di opportunità futura: la delega per la riforma del sistema di promozione dell'uso delle energie rinnovabili, per esempio, che si colloca al centro del progetto di transizione ecologica e in un punto focale rispetto al programma Next generation EU e al traguardo, ambizioso e giusto, della neutralità climatica al 2050; vi è poi la delega per il recepimento della direttiva sul *copyright*, che prevede maggiore attenzione alle garanzie dei prodotti delle aziende di comunicazione e dei singoli artisti, che spesso hanno visto negato il loro diritto di compenso nelle grandi multinazionali extraeuropee dello *streaming* e della diffusione. Si tratta di una direttiva di buon senso, su cui il mio Gruppo si è impegnato moltissimo e sulla cui necessità si è espresso anche il signor Mogol, che non è certo uno che non si intende dell'argomento. Nel testo che ci arriva dalla Camera c'è poi una modifica sostanziale relativa al recepimento della direttiva n. 343 del 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti giudiziari. È una modifica che avrà un immediato impatto sulla vita degli italiani e che, come primo risultato, dimostra chiaramente un netto cambio di passo verso il garantismo in questo Paese. un cambio di passo non solo a livello di politiche europee, ma anche rispetto agli aspetti giuridici che questo testo ci ha riconsegnato grazie al lavoro svolto dai colleghi di Forza Italia alla Camera relativo al rafforzamento della presunzione di innocenza e che ha visto il ministro Cartabia, che ovviamente ringraziamo, coerente con quella linea garantista che contraddistingue i sistemi democratici maturi. Tutto ciò è l'emblema di un cambiamento dell'assetto culturale del Paese, di una maturazione collettiva come classe politica che dovevamo da tempo ai nostri cittadini. La presunzione di innocenza e il diritto a un equo processo sono sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, per la maggior parte già accolti, come ha ricordato il collega Caliendo prima, nell'ordinamento giuspenalistico italiano. Eppure, recepire oggi la direttiva europea n. 343 del 2016 assume un significato estremamente importante di visione e costruzione collettiva. C'è un passaggio contenuto nel «considerando» 19 che, rapportato a ciò che spesso accade nel nostro Paese, assume una forte rilevanza emblematica. Lo cito testualmente. L'ha fatto prima che il collega Caliendo. «Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai *media*, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come colpevoli, fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata». Eppure spesso è cattiva prassi che indagati e imputati vengano presentati all'opinione pubblica come se fossero persone già condannate in via definitiva. Ogni giorno sono pieni i giornali di casi di indagati messi alla gogna e giudicati prima di un giusto processo. Questa modifica avvenuta alla Camera ci consente e, anzi, ci obbliga a una riflessione profonda sul perché, nonostante anche il nostro ordinamento punisca la diffusione di immagini che mostrano gli indagati come fossero già colpevoli, ci troviamo oggi quasi increduli, con gioia ovviamente, per il recepimento di una direttiva europea che va ulteriormente nella direzione di giustizia e civiltà. Questa sembra essere una di quelle volte in cui il «ce lo chiede l'Europa» ci può davvero portare un beneficio in termini di stato di diritto, un beneficio reale che riguardi tutti gli schieramenti politici e che faccia cessare quel costume tutto italiano del garantismo di facciata quando si parla di se stessi, alternato invece a uno spirito forcaiolo nell'accusare l'avversario, un atteggiamento che mi sento di dire con certezza - e verrà riconosciuto da tutti i colleghi in quest'Aula - Forza Italia non l'ha mai avuto. Sappiamo che il lavoro è ancora lungo e resta, ad esempio, urgente sollecitare la riforma in materia di aiuti di Stato e concorrenza, ormai del tutto distonici rispetto all'evoluzione delle relazioni commerciali internazionali. Comunque, è stato fatto molto con l'esame di questo provvedimento. Annuncio, pertanto, il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

far esprimere le Commissioni di entrambe le Camere, discutere in Assemblea di emendamenti e ordini del giorno e tornare ad avere nel Parlamento un organismo centrale della nostra democrazia. Sulla legge di delegazione è importante ribadire che nel suo primo passaggio in Senato è stato fatto un importante e approfondito lavoro in Commissione: tante audizioni, discussione su un gran numero di emendamenti e diverse modificazioni sostanziali del testo che abbiamo affrontato con uno spirito costruttivo, nonostante in quel momento storico ci si ritrovasse con una maggioranza diversa da quella attuale. Sono diversi gli aspetti che abbiamo cercato e, in alcuni casi, siamo riusciti a modificare; sono tutti afferenti a due tematiche che, se non affrontate in modo pragmatico, ma solamente ideologico, rischiano di arrecare ingenti danni al nostro settore produttivo. Mi riferisco al tema ambientale e a quello alimentare. Questa legge di delegazione è stata prodotta in un periodo pre-Covid, un periodo che risale a solo un anno fa e che ci sembra però lontanissimo per la portata disastrosa che tale virus e le conseguenti restrizioni ai movimenti, agli scambi e al commercio hanno causato sull'economia globale. All'interno di questo provvedimento alcuni articoli portano con sé una visione punitiva delle aziende che non si adeguano alle strettissime direttive in ambito ambientale e anche in ambito agroalimentare In un periodo all'interno del quale alcuni dei nostri principali *asset* strategici industriali pagano un prezzo altissimo in termini di perdita di fatturato e di *standard* occupazionali, noi dobbiamo iniziare a ragionare in modo completamente diverso, più pragmatico e meno ideologico. Dobbiamo ragionare ponendoci due quesiti. Primo: quello che stiamo approvando aiuta le nostre imprese? E soprattutto, secondo: quali sono i risvolti occupazionali di tali imposizioni? Sono positivi o negativi? Andiamo nel concreto sull'articolo 3. Ci siamo fortemente battuti per una maggiore attenzione a tutto il settore dell'agroalimentare; Ci siamo fortemente battuti per una maggiore attenzione a tutto il settore dell'agroalimentare; noi crediamo che, nella direttiva che si va a recepire con l'articolo 3, non vadano applicati i «considerando» 28 e 58, semplicemente perché crediamo che, applicando la direttiva senza escludere questi considerando, si rischia di andare a cagionare un danno al settore agroalimentare, andando a tacciare come rischiosi, in termini di salute, alcuni nostri prodotti tipici. In questo è evidente che dobbiamo trovare una posizione unita come Paese e non dividerci in termini partitici. È palese come questa sia una battaglia che alcuni Paesi europei conducono con il chiaro intento di danneggiare il nostro settore agroalimentare, che è un'eccellenza

preponderante all'interno del Ministero. Difendere le nostre eccellenze italiane però, come già detto, non può essere un qualcosa che ci divide o che varia in base alla collocazione di un Ministero. stesso approccio si deve avere sull'articolo 5 e, in generale, sulla tematica ambientale. Siamo tutti legati alla tutela dell'ambiente, ma un conto è farlo in termini pragmatici, con studi sull'impatto occupazionale di alcune politiche a medio e lungo termine, un altro è abbracciare un'ideologia *green* sulla base di orientamenti politici globali dai quali sembra non ci sia via di fuga. Quanto costerà ciò in termini di occupazione nel settore dell'*automotive*? La logica di introduzione in massa dell'auto elettrica, che in tanti si augurano diventi la logica mondiale, quanti posti di lavoro farà perdere in termini di produzione, di assistenza post vendita, di riparazione? Quanti di questi lavoratori potranno essere riassorbiti in altri settori? Parliamo di cambiamenti epocali, che possono portare alla perdita di milioni di posti di lavoro, anche solo nel nostro Paese. A fronte di questi numeri, è doveroso parlare di programmazione, di impatti occupazionali, di piani di riassorbimento della manodopera ed è doveroso farlo in concomitanza con i bei discorsi sulla tutela dell'ambiente. Solo così può avvenire una reale transizione verso un'economia sostenibile, sia dal punto di vista ambientale che da quello occupazionale. In conclusione, siamo contenti che alcuni dogmi legati all'Unione europea stiano cadendo uno a uno. Siamo stati il primo partito a denunciare le follie dell'austerità e vediamo con piacere che si è ricominciato a parlare di crescita, di PIL, di piani economici a lungo termine e che lo spauracchio del debito e le paure per lo *spread* siano almeno per il momento accantonate. Abbiamo parlato e denunciato per anni il rischio che l'Unione europea diventasse una sorta di mostro burocratico e vediamo con piacere, anche se non lo avremmo voluto, che siamo tutti concordi sull'incredibile pasticcio combinato dalla Commissione in fase di contrattazione e approvvigionamento dei vaccini, un argomento sul quale bisognerebbe aprire una lunga discussione, perché tali errori hanno avuto impatto sul nostro Paese, sia in termini di perdita di PIL che di vite umane e non possiamo né sottovalutarlo, né dimenticarlo. Concludo, ponendo dei temi che abbiamo evidenziato anche in prima lettura in sede di approvazione della legge di delegazione europea. Innanzitutto, c'è il tema degli appalti pubblici. Teniamo conto della procedura di infrazione n. 2273/2018 e delle difficoltà operative generate dal codice dei contratti pubblici e puntiamo ad adeguarci alle disposizioni della direttiva europea sugli appalti pubblici; semplifichiamo e revisioniamo realmente tale settore e puntiamo a far ripartire il Paese. della mobilità e delle infrastrutture. Adeguiamoci alle disposizioni del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti; realizziamo gli interventi infrastrutturali che servono al nostro Paese per risultare parte integrante di uno o più assi transeuropei di collegamento, come quello della Torino-Lione, Torino-Lione, che purtroppo è tornata alla ribalta nazionale per i violenti scontri che si sono svolti a San Didero la scorsa settimana e per il tentato omicidio che un gruppo di antagonisti ha cercato di mettere in atto, tendendo ad altezza uomo un cavo d'acciaio attraverso la Torino-Bardonecchia, potenzialmente letale per chiunque. Da piemontese auspico che il Governo nomini al più presto un commissario all'opera perché, solo ribadendo fermamente negli atti la volontà di completamento dell'infrastruttura, daremo un senso a tutti i sacrifici subiti dalla popolazione della Val di Susa, dagli agenti delle Forze dell'ordine e dagli operai del cantiere.

torniamo a parlare di legge di delegazione europea, anche se del 2019: siamo al 2021 e siamo ancora fermi. Sono già intervenuto in dichiarazione di voto il 29 ottobre scorso su questo stesso provvedimento. Da allora poco è cambiato nel testo l'altro ramo del Parlamento ha solamente aggiunto una direttiva ritenuta importante in materia di giustizia - ma molto è cambiato dal punto di vista politico. Abbiamo un nuovo Governo, una nuova maggioranza più ampia, ma anche alquanto disomogenea. Oggi, tuttavia, segniamo un altro punto nel percorso verso l'attuazione dell'idea di Paese che come MoVimento 5 Stelle abbiamo in mente e per cui i cittadini ci hanno premiato alle urne nel 2018. Con l'approvazione di questo disegno di legge, infatti, avviamo la procedura per il recepimento di un cospicuo pacchetto normativo che, come consuetudine per la legge di delegazione europea, riguarda svariati campi: ambiente, tecnologia, comunicazioni, *copyright*,transizione energetica, giustizia, tutti temi attualissimi, che si legano indissolubilmente con il Piano di ripresa e resilienza in corso di ultimazione da parte del Governo. Il recepimento di questa normativa in questo particolare contesto storico assume ancora maggiore importanza, in quanto va a creare l'ambiente, l'*humus* normativo entro il quale il PNRR dovrà inserirsi e dispiegare tutte le potenzialità di rilancio e innovazione di cui il Paese ha bisogno. Per questo motivo il disegno di legge, pensato prima della pandemia, ha avuto nel corso dei passaggi parlamentari numerosissime modifiche con l'inserimento di ulteriori criteri di delega proprio al fine di instradare e controllare la nostra idea di rilancio e di sviluppo.

fatto nel corso della sua esperienza al Mise *(Applausi)* - con particolare riferimento alle comunità energetiche, che - lo ricordo - sono il frutto di una nostra lotta durata anni, sia nel Parlamento europeo che nel Parlamento italiano, e che abbiamo già tramutato in realtà, anticipando anche la direttiva comunitaria stessa. Penso poi alla direttiva sulla plastica monouso, su cui vorrei spendere alcune riflessioni. In quest'ultimo anno abbiamo assistito - lo dico con grande rammarico - a un notevole ricorso alla plastica monouso: un deciso passo indietro nel percorso virtuoso che si era innescato, dovuto alle nuove necessità manifestatesi a causa della pandemia in corso. Oggi, tuttavia, in un'ottica di rilancio e cambiamento, è opportuno riprendere la strada che avevamo intrapreso, abbandonando la plastica monouso e, al contempo, tutelando un comparto che vede l'Italia protagonista a livello europeo. Per questo motivo, voglio ricordare che in prima lettura è stato approvato un emendamento fortemente voluto dall'allora maggioranza, volto a chiarire la lettera della direttiva in modo da scongiurare un possibile erroneo recepimento che avrebbe causato ingenti danni ai nostri produttori, che invece devono essere accompagnati nella transizione verso produzioni e consumi maggiormente in linea con gli obiettivi ambientali che ci prefiggiamo. Penso inoltre al codice delle comunicazioni elettroniche inserito in questo disegno di legge di delegazione europea, fondamentale per lo sviluppo di una rete potente ed affidabile, nonché necessario per supportare il processo di digitalizzazione del Paese previsto nel PNRR e senza il quale lo stesso non potrebbe concretizzarsi al meglio.

con l'approvazione di oggi abbiamo la chiusura o scongiuriamo l'apertura di una serie di procedure di infrazione per mancato recepimento della normativa europea, procedure che pesano su una finanza pubblica già provata dagli sforzi fatti o che stiamo facendo per limitare il più possibile i danni causati dalla pandemia globale. Sono otto le procedure di infrazione su cui interveniamo, cui si sommeranno quelle della legge europea il cui esame è appena iniziato nella 14a Commissione del Senato. Infine, vorrei concentrarmi sulla linearità dell'azione del MoVimento 5 Stelle nelle maggioranze che hanno sostenuto i Governi Conte I e II prima, e Draghi ora. Sono cambiati tre Governi dall'inizio della legislatura e tuttavia il MoVimento 5 Stelle, grazie alla determinazione con cui persegue quell'idea di futuro che abbiamo in mente da ormai un decennio, è sempre riuscito ad incidere e ad indirizzare l'azione di Governo perché mettesse in pratica quanto avevamo proposto agli elettori nel 2018. Anche se è intervenuta la pandemia, da tre anni, con la nostra azione di Governo nei due rami del Parlamento gettiamo le basi per un'Italia migliore e pronta ad attuare quei necessari e non più rimandabili cambi di marcia che ci consentiranno di uscire dalla lentezza, se non dall'immobilismo, che ha contraddistinto lo sviluppo negli ultimi decenni, e dare un nuovo slancio per una crescita in linea con i nostri *competitor* internazionali. Certo, oggi una maggioranza così ampia e variegata complica un po' le cose. Tuttavia, il MoVimento 5 Stelle, come promesso, dando la fiducia a questo Governo, vigila e vigilerà sempre attentamente ed è pronto a segnalare ogni deviazione eventuale da quanto concordato in sede di formazione dell'attuale Esecutivo. A tal proposito, mi permetto di segnalare che le Camere ancora attendono di poter visionare il Piano nazionale di ripresa e resilienza definitivo, anche se capiamo che il tempo è poco, seppure l'attuale Governo abbia potuto giovarsi del grande lavoro fatto dal Governo Conte II. I rappresentanti dei cittadini, cioè noi, eletti dagli stessi, non possono essere lasciati all'oscuro e senza possibilità di intervenire sui contenuti di un Piano che segnerà l'Italia almeno per i prossimi venti So che a breve, la prossima settimana, il Presidente del Consiglio verrà in Aula per riferire sul tema, ma credo fermamente che sarebbe estremamente importante non solo per il Parlamento, ma per il Paese, poter visionare in anticipo i progetti contenuti nel Piano per dare il nostro fattivo contributo.

la struttura del Senato della Repubblica che ci permette di lavorare in maniera puntuale e attenta. *(Applausi)*.

lo Stato Italiano a pagare i debiti della pubblica amministrazione con puntualità, questo pagamento dei debiti non avviene e spesso mette in difficoltà le piccole imprese che operano in relazione con Tante volte, però, la pubblica amministrazione si ritrova a dover fare i conti con un'Europa che chiede cose che vanno a smantellare il sistema e la tipicità italiana. Penso ad esempio al caso Tercas: qui l'Europa ha messo le proprie impronte digitali sull'affossamento del nostro peculiare sistema bancario, quello di banche legate al territorio, e non ha solo commesso l'errore in prima battuta, ma ha anche fatto ricorso e perso. Il caso Tercas è stato un po' il paradigma che ha portato all'affossamento all'affossamento di un sistema bancario molto peculiare. Poi l'Europa, mai come in questo tempo di emergenza Covid, proprio sull'emergenza vaccinale ha replicato gli stessi commessi, in prima battuta, di fronte alle prime avvisaglie dell'emergenza, senza dotarsi di un protocollo comune, di un linguaggio comune e di un sistema di osservazione comune che potessero dare delle indicazioni ai Paesi dell'Eurozona e dell'Unione europea. Penso anche a quanto succede rispetto al tema della concorrenza. Non ho capito che fine Non ho capito che fine abbia fatto la lettera che la Vestager, commissario europeo alla concorrenza, ha inviato al nostro Governo rispetto ai porti italiani. Non vorrei che corressimo il rischio di trovarci di fronte ad una progressiva e silenziosa lettera la Vestager l'ha scritta alcuni mesi orsono, ma da parte del Governo non abbiamo ancora capito che tipo di risposta abbiate dato, perché tra l'altro va ad incidere sulla parte fiscale della gestione dei porti. Delegare continuamente all'Europa rischia di essere una delega in bianco che smonta progressivamente l'Italia, l'italianità e il *made in Italy.* Andate a chiedere alla comunità dei pescatori quanto bene facciano tutte queste normative europee che appesantiscono in termini burocratici l'attività della pesca o l'attività dell'agricoltura. Ovviamente per Italexit il voto non può che essere contrario e ringrazio ancora l'Assemblea per l'attenzione.

**Il Senato approva.**

fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; *b)* Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. Art. 2. **Approvato**

che ormai sono datati al 2002 e al 2006, quasi tutti recepiti dalla normativa nazionale in materia di lavoro dignitoso e produttivo e di sicurezza sui luoghi del lavoro. quindi, a compimento una ratifica quasi scontata. L'intento è che questi documenti internazionali contribuiscano a a costruire la cultura per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e a creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre mediante un'azione progressiva e coordinata sia a livello nazionale che di impresa, con la piena partecipazione di tutte le parti interessate. In particolare, tali norme internazionali mirano a costituire un quadro di riferimento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione delle funzioni e delle responsabilità dei vari attori, l'approfondimento della conoscenza delle questioni della sicurezza sul lavoro, come dicevo già ampiamente recepito da molta parte della normativa italiana. L'analisi delle compatibilità dell'intervento di ratifica non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell'Unione europea e con gli obblighi internazionali. Si propone quindi l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare l'Accordo tra l'Italia e l'Ecuador, sottoscritto nel luglio 2016, in materia di cooperazione di polizia, che sancisce l'impegno dei due Paesi ad intensificare la collaborazione bilaterale per prevenire, contrastare e condurre indagini sulla criminalità nelle sue varie forme, ponendosi quale strumento giuridico per regolamentare la cooperazione di polizia sotto il profilo strategico ed operativo. In particolare, l'Accordo indica i settori della cooperazione bilaterale relativi al crimine organizzato transnazionale, alla tratta di esseri umani, ai traffici di stupefacenti, di migranti, di armi e di beni culturali; alla ricerca dei latitanti, al riciclaggio e alla criminalità informativa. Il disegno di legge si compone di quattro articoli e l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale,

tutti strumenti giuridici adottati nell'ambito delle Nazioni Unite. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Signor Presidente, sarò estremamente veloce. Tale Accordo intende fornire un quadro giuridico essenziale per l'approfondimento della disciplina dei rapporti tra l'Italia e l'Afghanistan in questioni molto importanti che riguardano l'innovazione, l'istruzione e la formazione. Cooperazione oggi più che mai fondamentale, anche in funzione della necessità di continuare a fornire supporto supporto al popolo afghano in seguito al ritiro delle truppe Nato dal territorio. L'annuncio della prossima conclusione della missione alleata è stata accolta con favore e grande entusiasmo. Tuttavia deve necessariamente essere accompagnata da iniziative di cooperazione allo sviluppo ed attività volte alla maggior tutela dei diritti umani della popolazione civile, per evitare che lo spazio lasciato dalle truppe occidentali sia riempito da nuovi conflitti intestini. L'Italia è storicamente impegnata nel sostegno allo sviluppo dell'Afghanistan; ne sono un esempio gli accordi con il nostro Paese, che contribuisce a offrire supporto alle piccole imprese, all'agricoltura ai mercati rurali o la riabilitazione di strade o corridoi. L'intesa che ci troviamo oggi ad esaminare esplicita innanzitutto l'impegno delle parti a sviluppare attività che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, a a promuovere i rispettivi patrimoni culturali, a rafforzare la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a promuovere programmi multilaterali, nonché la diffusione delle rispettive lingue e culture, a favorire la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi e ad incoraggiare la collaborazione tra le rispettive università e istituti di formazione superiore. Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

culturale, scientifica e tecnologica tra l'Italia e il Governo della Repubblica dell'Afghanistan. Non sfuggirà ai nostri colleghi il fatto che questo Accordo arriva a seguito del ritiro delle truppe dal suolo afgano. afgano. Tale decisione che fu presa inizialmente nel febbraio 2020 dall'Amministrazione statunitense di Trump, poi confermata nei fatti nel settembre 2020, ha trovato seguito in questi giorni perché la nuova amministrazione, sebbene sia stata annunciata come completamente differente, in realtà ha seguito il solco tracciato dall'Amministrazione Trump. Tanto che l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di trovare meravigliosa e positiva la decisione dell'Amministrazione Biden. quindi che si stia avviando una nuova epoca per l'Afghanistan e l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica al nostro esame cade proprio a proposito. Pertanto, nell'esprimere il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, esprimo anche apprezzamento per l'Amministrazione prima Trump, poi Biden, che hanno il merito di aver deciso di ritirare finalmente le truppe dall'Afghanistan.

nel febbraio 2018, intende porsi quale strumento regolatore del trasporto di persone e merci su strada tra l'Italia e la Tunisia, per agevolare lo sviluppo dell'interscambio commerciale e della mobilità tra i due Paesi.

l'Assemblea è chiamata ad esaminare il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Bolivia in materia di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nel marzo 2010. Tale Accordo, destinato a sostituire una precedente intesa di settore, risalente al 1953, esplicita innanzitutto l'impegno delle parti a promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue e culture e a favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei. L'Accordo impegna inoltre le parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e dell'ambito radiotelevisivo, nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta in 179.180 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e in 188.300 euro annui a decorrere del 2023, nonché in ulteriori 78.840 euro, a decorrere dall'anno 2021. Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

rappresentanti del Governo, colleghi, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge, già approvato alla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritto dall'Italia e dal Governo della Repubblica del Kosovo nell'aprile del 2019. Come si evince dalla relazione introduttiva al disegno di legge, la scelta di disciplinare la materia attraverso un'apposita convenzione bilaterale è stata dettata dalla mancanza di altri strumenti giuridici applicabili al caso, non avendo il Kosovo aderito alla Convenzione del marzo del 1993 del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate. L'Accordo è finalizzato a consentire il trasferimento - nel proprio Stato - dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo da permettere di scontare la pena loro irrogata a seguito di sentenza di condanna irrevocabile nel proprio Paese di origine. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li valuta complessivamente in euro 5.114 5.114 annui a decorrere dal 2020, ascrivibili essenzialmente alle spese per il trasferimento delle persone condannate e per le missioni dei loro accompagnatori. L'analisi della compatibilità dell'intervento non segnala criticità di ordine costituzionale né di contrasto con la normativa dell'Unione europea o con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali. Il Protocollo, firmato il 16 novembre 2009, rappresenta il culmine di oltre vent'anni di lavoro a livello intergovernativo in seno al Consiglio d'Europa in tema di partecipazione democratica a livello locale, iniziato con la firma della Carta europea delle autonomie locali. Il documento, approvato nel 1985 in seno al Consiglio d'Europa e ratificato ad oggi da tutti e 47 i Paesi membri dell'organismo continentale, obbliga le parti ad applicare le regole fondamentali per garantire l'indipendenza politica, amministrativa e finanziaria degli enti locali, prevedendo che il principio dell'autonomia locale sia riconosciuto dal diritto nazionale e protetto dalla Costituzione, permettendo così agli enti locali di essere eletti con suffragio universale. Il Protocollo addizionale, la cui ratifica è oggi al nostro esame, prevede che alla Carta europea delle autonomie locali sia aggiunta anche un'altra dimensione, relativa al diritto della persona a partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali, ovvero il diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze e delle responsabilità dell'autorità locale. L'articolo 3 del disegno di legge, nel porre una clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

vorrei fare un brevissimo inciso su questo Accordo, che è molto interessante. Sebbene sia datato al 1985, arriva in Aula in questi giorni.

di chiunque a partecipare agli affari di una collettività locale. Evidenzio particolarmente questo aspetto, perché credo sia interessante lasciare agli atti ciò che è accaduto oggi in Commissione affari esteri: abbiamo audito l'ambasciatore cinese, il quale, sollecitato in maniera molto importante da svariati commissari, tra i quali il sottoscritto per la Lega, ma anche da altri colleghi del centrodestra, è stato incalzato fortemente sul tema dei diritti umani. Sostanzialmente, ci ha risposto che chi non è d'accordo con le direttive del Governo non può esercitare un ruolo

un tema sul quale dobbiamo riflettere per decidere quale sia l'atteggiamento da tenere. Da una parte, stiamo parlando del diritto di tutti a partecipare alla vita politica delle comunità, a prescindere dall'indirizzo

intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, ringraziando il relatore Aimi per il lavoro svolto. Spero che, una volta ratificato questo Accordo, potremo finalmente cambiare una legge assurda, che impedisce ad alcune comunità locali italiane di partecipare alla vita delle proprie amministrazioni locali, come nel caso di coloro che abitano nei Comuni non capoluogo di Provincia delle cosiddette Città metropolitane, che si vedono eleggere il sindaco metropolitano da altri, ossia da coloro che abitano nel capoluogo. Spero che con l'Accordo internazionale saremo spinti a cambiare una legge assolutamente assurda e incoerente con i principi democratici.

rappresenta una convenienza reciproca per entrambe. La Tunisia è un Paese strategico per gli interessi nazionali italiani

elettrica atta all'interscambio di energia tra l'Italia (e, quindi, l'Europa) e il Nord Africa. L'Accordo è stato sottoscritto dai due Paesi il 30 aprile 2019. È un progetto ambizioso per la realizzazione e gli sviluppi futuri. mi sembra doveroso sottolineare il significativo valore strategico, come ha già ricordato il relatore, e geopolitico dell'opera, che riposiziona il nostro Paese nello scacchiere politico nordafricano. L'opera, nella proposta per l'energia e il clima della Commissione europea, si pone come obiettivo l'integrazione della Tunisia e dell'intera regione nel mercato europeo. Questa brevissima introduzione si rende necessaria per meglio far comprendere l'importanza strategica: ovvero allargare il mercato energetico e delle fonti rinnovabili a milioni di persone. L'opera di cui parliamo prevede la realizzazione messa in

atti quale sia stato il nostro intervento in Commissione su questo Accordo, perché durante la discussione è emerso, anche dalla relazione presentata da Terna, che questo investimento, che non è a costo zero (a parte la componente (a parte la componente europea, c'è un investimento anche da parte italiana), avrebbe avuto un riflesso sulla bolletta degli italiani. Chiaramente il Gruppo Lega si è immediatamente attivato e abbiamo chiesto un approfondimento al Governo. Questi approfondimenti sono arrivati e il e il Garante ha rassicurato sul fatto che dal 2026 gli aumenti saranno sostanzialmente minimi. Volevo lasciare agli atti questo intervento, perché secondo me è stato molto significativo. Esprimo in questa sede il voto favorevole del Gruppo Lega.

consegnerò la relazione, limitandomi a sottolineare come la Svizzera, che è Paese membro dell'ESA (l'Agenzia spaziale europea), abbia un ruolo importante all'interno del programma Galileo, in termini di servizi tecnologici e logistici. Si rendeva pertanto necessario andare a ratificare l'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, per rafforzare la cooperazione in questo ambito. L'articolo 3 del disegno di legge pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri. Per il resto, chiedo

intervengo sul video veramente scandaloso e vergognoso di ieri di Beppe Grillo.

perché mi volevo rivolgere anche ai colleghi e, in modo particolare, alle colleghe del MoVimento 5 Stelle.

e che in qualche modo è stata fatta passare per colpevole.

giudicando se quei ragazzi sono colpevoli o innocenti, perché per questo c'è la magistratura e noi crediamo nella magistratura. Siamo però garantisti e, soprattutto, non ci possono essere momenti

un conto è difendere i valori della giustizia, un conto è il giustizialismo e un conto sono la spettacolarizzazione e l'aver deriso e ridicolizzato il dolore e la sofferenza di una ragazza e della sua famiglia. Non solo Non solo dunque chiediamo le scuse di Beppe Grillo a quella ragazza e a quella famiglia, ma chiediamo anche le sue scuse in quanto personaggio pubblico, che ha utilizzato il suo potere mediatico per

cercare forse il silenzio e non dire una parola su questa vicenda. Secondo me, signor Presidente, sarebbe stato meglio non esprimersi in questo senso. Ha deciso però, ancora una volta, di far prevalere il giustizialismo e la spettacolarizzazione

e, soprattutto, dignità per tutte le donne *(Applausi)*, perché con quel video sono state offese tutte le donne e, prima di tutto, coloro che hanno subito violenza.

C'era una volta un partito che inveiva contro tutti: ero Vice Presidente del Senato, usai a sproposito il termine "*handicap*", "handicappato", che oggi è politicamente scorretto e non va usato - oggi si usano termini diversi per indicare una difficoltà fisica e personale e una senatrice, che oggi non siede più sui banchi del Gruppo MoVimento 5 Stelle, chiese le mie dimissioni, perché avevo sbagliato. Mi scusai, presiedendo i lavori, perché avevo sbagliato a usare una parola che venti o trent'anni fa era nel gergo e oggi è considerata un'offesa. È vero che Grillo non è un parlamentare e che non sta in quest'Aula, però ha deciso Governi e non Governi; qui ci sono colleghi che non avrebbero votato alcuni Governi, se Grillo non glielo avesse ordinato, quindi è un capo politico a tutti gli effetti *(Applausi)*, un *leader* che decide della democrazia italiana. Peraltro, ai partiti ancora credo, quindi, se un partito decide una linea, è anche giusto che poi un parlamentare esegua. E Grillo è intervenuto nel dibattito politico. politico. Parlo dai banchi di un partito ipergarantista, Forza Italia, che ha brandito il tema della giustizia in tutti i momenti, spesso incompreso e dileggiato, soprattutto da Grillo e dal suo MoVimento, che ha invocato la forca in ogni caso, ma non per il proprio figliolino. Essendo garantisti, auguriamo a suo figlio di essere liberato dalle accuse - che poi non sono state ancora formalizzate e non mi pare che ci sia ancora il rinvio a giudizio - però Grillo con questo linguaggio, i gesti e le parole che ha usato ha messo una lapide sulla sua rivoluzione morale. Era più bravo quando faceva la pubblicità dello yogurt, perché allora almeno faceva ridere

perché perfino nelle mura domestiche non hanno il coraggio, la possibilità o l'agibilità - non so quale termine usare, ditelo voi - di telefonare a una caserma o a un commissariato perché minacciate. L'abbiamo discusso in Parlamento e abbiamo fatto leggi: abbiamo introdotto il reato di *stalking* e quant'altro. Non so come siano andati i fatti e mi pare strano che Grillo dica di avere il video: che ci fa con questo video? Vada alla procura e lo consegni. Quanto alla vicenda sessuale col video fatto, è vero che c'era una Presidente di Commissione che aveva riempito la casa di telecamere. Ci siamo scordati questo episodio di qualche tempo fa:

rispetto per le istituzioni e l'autodifesa, perché era suo figlio. Rispetti la verità, rispetti le donne e rispetti la magistratura. Ci ha insegnato cose che non conosceva neanche lui, torni a pubblicizzare lo yogurt.

«Vile, tu uccidi un uomo morto». Non sono questo, come Grillo non è certamente Ferrucci. Credo che abbia grandissime responsabilità: non voglio ricordare in quest'Aula

Il suo contenuto principe era proprio l'utilizzo della magistratura, di quell'essere giacobino che certamente bene a questa Nazione non ha fatto. Prendo atto di questo cambio repentino di Grillo e vi devo dire che, da madre, lo comprendo; l'amore per un figlio è così grande essere riuscito a incidere sul credo di Beppe Grillo di tutti questi anni. L'amore di un figlio ha fatto capire un'altra cosa, perché - ce lo dobbiamo dire, colleghi, con chiarezza - questo tipo di giustizia è come un cancro: quando non si prova sulla propria pelle, non si capisce la devastazione che procura. È la stessa cosa, colleghi, quando arrivano queste bombe di giudizi sommari o, peggio, di pregiudizi all'interno delle famiglie. Grillo adesso sta capendo

ma soltanto colui che era nemmeno indagato, ma soltanto sospettato. E Grillo già faceva sentire il tintinnio delle manette. Caro Grillo (mi rivolgo a lui), da mamma ti capisco, perché ognuno di noi per difendere il proprio figlio sarebbe pronto a farsi uccidere. Attraverso questo cambio repentino devo

chi di spada ferisce, di spada perisce. Grillo, hai invocato tante volte questa giustizia piena di pregiudizi e questa volta ce l'hai in casa: mi dispiace, ma devi fartene una ragione.

donne su dieci, però, non riescono a denunciare. C'è troppa urgenza di intervenire, per questo dovevamo approvare al più presto la nostra proposta sul codice rosso e le norme antiviolenza su donne e bambini»; «abbiamo previsto pene più forti per chi si macchia di reati così gravi». E ancora: «Il MoVimento 5 Stelle ha voluto inserire anche la norma che allunga i tempi per denunciare l'aggressione per fatti di violenza: non più sei, ma dodici mesi. Un passo così importante è delicato e ha bisogno del tempo necessario per maturare». Questo articolo

l'avete scritto. L'ha scritto e l'ha condiviso sicuramente il vostro *leader*. Non entro nel merito di come si comporta, ci mancherebbe altro; lo guardo come uomo e oggi quest'uomo ha reso vergogna all'Italia. *(Applausi)*. In quest'Aula spesso portiamo quello che succede in casa degli altri. Parliamo delle donne maltrattate, violentate o sequestrate in casa degli altri e facciamo discussioni per ore e ore. Oggi invece dobbiamo guardare in casa nostra, perché abbiamo reso l'Italia piccola e barbara,

il reato consumato al momento, ma ci sono le conseguenze che si porterà dietro per una vita. Ha in qualche maniera dileggiato le donne e reso vano il lavoro che il Senato

madre e tanti qui sono genitori. A volte i genitori devono insegnare ai loro figli cos'è il bene e cos'è il male e tante volte sbagliano e devono attendere. Al signor Grillo posso solo dire che avrebbe fatto bene a tacere *(Applausi)*, perché a volte anche

ma con un fatto importante. L'ennesimo sequestro di uno scarico abusivo illecito, ritrovato ad Acerra, con sversamento nelle acque reflue dei Regi Lagni, richiama ancora una volta di più l'attenzione sulla gravissima situazione degli sversamenti incontrollati di rifiuti speciali riversati abusivamente nell'ambiente e, nel caso specifico, nella serie di canali che si diramano nel territorio della periferia a Nord-Est di Napoli e nella parte meridionale della provincia di Caserta, che costituiscono e rientrano nel sistema dei Regi Lagni. Tutti i veri e propri delitti e scempi ambientali che continuano costantemente a verificarsi in questi territori, in cui - non dimentichiamolo - è localizzata la cosiddetta terra dei fuochi, devastano le nostre terre, avvelenano le nostre acque e inquinano i nostri territori. Gli smaltimenti illeciti insistono sui nostri territori, incuranti delle grida di dolore che si levano da ogni parte ogni giorno e delle gravissime e colpevoli conseguenze del disastro ambientale che stanno provocando. Essi rappresentano una delle dimostrazioni più abiette del punto di non ritorno cui sono arrivate la bramosia umana e l'assenza di senso di responsabilità e di appartenenza di alcuni personaggi, che potremmo definire vere belve, che, oltraggiando la legge, non si fermano nemmeno davanti alle tante vittime che i veleni da essi scaricati senza controllo purtroppo provocano, in un'*escalation* incontrollabile, con un rapporto causale ormai dimostrato, senza ombra di dubbio, con le patologie più varie, *in primis* quelle tumorali, che colpiscono la nostra comunità, senza risparmiare nessuna fascia d'età. Nonostante le attività di contrasto ai reati ambientali da parte dei Carabinieri, e in particolare dei forestali, proseguono senza sosta questi scempi ambientali, continuano con cadenza periodica e non si riescono realmente a fermare. Pneumatici, materiali plastici e ferrosi, guaine, liquidi inquinanti, materiali di risulta, residui provenienti da concerie e tutta una serie di rifiuti speciali vengono accantonati e smaltiti abusivamente senza precauzioni e senza rispettare le modalità previste dalla legge. Il risultato finale è che si avvelenano i nostri territori. Un reato commesso contro l'ambiente in cui viviamo è un delitto commesso verso il nostro futuro e i nostri figli. *(Applausi)*. c'è un altro video che gira in questi giorni a cura del sito www.notav.info sui responsabili di lanci ad altezza uomo. Si vedono e si sentono chiaramente uomini delle Forze dell'ordine e dell'Arma dei carabinieri in tenuta antisommossa, in un'area boscosa dietro una staccionata, sparare ripetutamente lacrimogeni ad altezza uomo, di notte, verso una piana da cui provengono canti.

prodotto due emorragie cerebrali e plurime fratture al volto. PRESIDENTE. Senatrice, lei riferisce fatti di cui ha conoscenza diretta? È stata ferita durante un'azione di sgombero in Val di Susa, un'azione spropositata delle Forze dell'ordine. Non ci sono più parole per descrivere quanto sta avvenendo in Val di Susa, una vera e propria occupazione militare del territorio, si legge sul sito. Non possiamo continuare a fingere di non sapere e di non vedere che i decreti-legge su immigrazione e sicurezza, che non sono stati modificati per la parte sicurezza, sono la base di questi inasprimenti e dei tanti fermi e arresti nel Paese, in una crescente compressione dei diritti costituzionali, aggravata